Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario della settimana corrente e il nuovo calendario dei lavori della prossima settimana fino al 26 febbraio. Nel corso di questa settimana - possibilmente entro la seduta pomeridiana di domani - saranno discussi, oltre ai provvedimenti all'ordine del giorno di oggi (decreto-legge sulla semplificazione normativa e modifica alla legge elettorale per il Parlamento europeo), i decreti-legge recanti proroga di missioni internazionali e disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni e *referendum*. Per tutti i provvedimenti previsti dal calendario di questa settimana si è proceduto alla ripartizione proporzionale dei tempi, ferme restando eventuali cessioni concordate tra i Gruppi. Nella seduta antimeridiana dì giovedì 19 febbraio saranno esaminati i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e due ratifiche di accordi internazionali, con la Federazione Russa in tema di cooperazione alla lotta alla criminalità e con gli Stati Uniti in materia di doppie imposizioni. Nella seduta pomeridiana di giovedì 19 si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata, con trasmissione diretta televisiva della durata di un'ora, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su questioni relative alle condizioni di rischio sull'autostrada Salerno - Reggio Calabria, nonché alla privatizzazione della società Tirrenia e ai collegamenti con le isole, salva la disponibilità del Ministro a rispondere ad altri quesiti su materie di sua competenza. Il calendario della prossima settimana prevede, a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 24 febbraio, l'esame del disegno di legge collegato in materia di semplificazione, competitività e processo civile, nonché - ove concluso dalla Commissione - del disegno di legge collegato sulla produttività del lavoro pubblico. Nella seduta antimeridiana di giovedì 26 febbraio saranno inoltre discusse mozioni sulla crisi dei mercati finanziari. La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito che l'inizio dell'esame dei disegni di legge in materia di testamento biologico abbia luogo in Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana di giovedì 5 marzo, nel testo definito dalla Commissione o nel testo base del relatore. Infine, sono stati indicati come prioritari tra gli argomenti delle prossime settimane il disegno di legge collegato in materia di internazionalizzazione imprese ed energia e il disegno di legge comunitaria 2008.

«La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. Esprime, poi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2 e 1.3. Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti». di semplificazione normativa, anche in relazione al particolare rigore con il quale deve essere valutata la corrispondenza al testo di emendamenti presentati a provvedimenti di urgenza. Pertanto, ai sensi dell'articolo 97, comma primo, del Regolamento è improponibile l'emendamento 2.0.1.

simile se non identico all'ordine del giorno approvato dalla Commissione; c'è una differenza, però, al secondo capoverso del dispositivo,

Diciamo così: potrebbe sembrare un'insistenza persecutoria, quella di proporre un emendamento abrogativo della legge Alfano, una legge diventata tale nel 23 luglio 2008, ma, in realtà, la notizia di oggi

e per il quale è stata chiesta e data una condanna a quattro anni e sei mesi, dimostra che c'è stato un processo per corruzione in cui l'avvocato Mills era imputato di essere corrotto dall'azienda del Presidente del Consiglio. Lui é stato condannato. Se lui é stato condannato, qualcuno lo ha corrotto. Allora, la richiesta di abrogare la cosiddetta legge Alfano viene rafforzata da una questione di attualità. Noi abbiamo un Presidente del Consiglio la cui azienda ha corrotto l'avvocato Mills e non si può fare niente su questo, perché il Presidente del Consiglio è protetto da una legge che sancisce la fine dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge - soprattutto della sua: della sua: sciolto dal vincolo delle leggi noi dobbiamo assistere impotenti a questo stato di cose. Capisco che in questo contesto sia inammissibile un emendamento che richiede l'abrogazione della legge Alfano, però voglio mettere agli atti che la pura e semplice realtà giudiziaria esistente nel Paese testimonia che quella legge è ingiusta e che nella realtà in cui viviamo è impossibile procedere contro chi, come attestato da questa condanna, ha corrotto l'imputato in questione. Sarà poco elegante insistere su argomenti di questo tipo, ma purtroppo è la nostra stessa situazione istituzionale che non è elegante.

Senatore Pastore, non è obbligatorio citare termini inglesi. Ci troviamo più a nostro agio con l'italiano.

con le Regioni e mira a rendere più chiaro quanto previsto nel decreto‑legge, soprattutto nella parte modificata dalla Camera. Naturalmente sono disponibile a una riscrittura se il Governo ritenesse di dover meglio precisare qualche passaggio.

che sicuramente verrà preso in considerazione rispetto al progetto «Normattiva». Se dovessi però introdurre per legge l'individuazione dello specifico soggetto, in fase di trattativa, rispetto al costo dell'operazione, perderei qualsiasi tipo di margine di manovra. Da oggi siamo scesi di quasi un milione rispetto al prezzo inizialmente richiesto; intendo proseguire con questa trattativa spendendo il meno possibile e, quindi, invito i presentatori al ritiro

del giorno G1.101, a condizione che vengano espunte le ultime parole "ferma restando la prosecuzione dei finanziamenti regionali per la banca dati in essere", proprio per non andare a toccare l'autonomia finanziaria delle Regioni.

ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400». La motivazione è tecnica, ma ha il suo peso. Il comma 2 dell'articolo 2

non precisa però la natura giuridica di tale atto. Sembra presumibile - ma solo presumibile - che esso debba essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica per poter procedere all'abrogazione di atti ad esso equiordinati, come i regolamenti governativi. Il presente emendamento, quindi, rende esplicita e chiarisce la natura regolamentare degli atti, prevedendo la loro adozione ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, numero 400. numero 400. In un decreto‑legge sulla semplificazione normativa ci si aspetta legittimamente una certa chiarezza normativa dal Governo.

regolamenti che individuino i regolamenti abrogati per effetto delle varie situazioni in evoluzione. Quindi, anche queste disposizioni contenute nel

del relatore. Anch'io sollecito il senatore Pardi alla trasformazione del suo emendamento in un ordine del giorno che possa puntualizzare un aspetto che veniva

e questa norma potrà essere ripescata con i decreti legislativi di cui parlava prima il Ministro. Pertanto, invito al ritiro per coerenza con quanto detto precedentemente.

e si appresta a farlo anche qui al Senato. Non sto a riportare alla memoria le osservazioni critiche già svolte dal collega Mascitelli. Tengo soltanto a ribadire che gli elementi della semplificazione legislativa non stanno soltanto in questo provvedimento:

Non vorrei che sulla questione della semplificazione legislativa si creasse una sorta di fenomenologia dello spirito diffuso, per cui si possono ritrovare elementi di semplificazione sparsi ovunque,

proprio perché la necessità della semplificazione legislativa ha un fondamento, mi sembra motivo di

rigoroso mantenere un filone unico afferente al resto del corpo legislativo, per evitare questo gioco di domanda e risposta che le leggi alla fine fanno tra loro.

una sua inevitabile ragion d'essere data la difficoltà, però, l'intervento qui è rivolto a richiedere una reale applicazione dello spirito della semplificazione.

Presidente, la semplificazione e la riduzione dello *stock* legislativo, avviato con l'articolo 24 del decreto-legge n. manovra d'estate), e perfezionato con il decreto-legge in discussione tramite l'espressa abrogazione di tutti quegli atti di cui si ritiene cessata la vigenza, è un primo passo nella direzione di una profonda revisione del *corpus* normativo del nostro Paese, che è condiviso e valutato positivamente dal Movimento per l'Autonomia, nel quadro di un'organica riforma, a partire dalla redazione di testi unici, dalla riduzione della proliferazione legislativa e da una attenta revisione delle modalità di redazione dei testi normativi, troppo spesso farraginosi e contorti e non di rado di difficile interpretazione. L'ampiezza dell'intervento abrogativo operata con la manovra d'estate ha determinato, inevitabilmente, l'abrogazione di alcune norme ancora necessarie, la cui vigenza non è ancora interamente cessata ed i cui effetti sui cittadini meritavano forse una più approfondita valutazione. La disposizione contenuta all'articolo 3 del decreto-legge al nostro esame corregge queste sviste, consentendo di sottrarre all'effetto abrogativo *de quo* gli atti normativi per i quali le amministrazioni competenti hanno ritenuto indispensabile il mantenimento in vigore. Tra queste norme vi sono due disposizioni che, negli anni, hanno regolato le procedure di erogazione dei contributi statali per la ricostruzione dei territori del Belice danneggiati dal sisma del gennaio 1968: la legge n. 464 del 1978 e la legge n. 433 del 1991, elencate all'allegato A rispettivamente alle voci 2990 e 3309, che vengono salvate dall'abrogazione anche per la sensibilità del Ministro Calderoli, che in questa sede ringraziamo. Si tratta di disposizioni che, regolando le procedure giuridiche e tecnico-amministrative e consentendo l'erogazione delle risorse finanziarie stanziate dalla legge finanziaria 2007 e appostate in bilancio a legislazione vigente, rappresentano lo strumento giuridico essenziale per il completamento degli interventi di ricostruzione dell'edilizia privata. In particolare, la legge n. 464 contiene le norme generali che presiedono al riconoscimento del diritto al contributo, alla quantificazione delle provvidenze economiche ed alla loro erogazione, nonché alle procedure di approvazione dei progetti attraverso il funzionamento di una commissione. La legge n. 433 del 1991 contiene invece disposizioni che regolano l'acquisizione al patrimonio dei Comuni delle aree o degli immobili di risulta per i quali i cittadini hanno ottenuto il contributo di ricostruzione in un nuovo sito, consentendo ai Comuni stessi di intervenire per la salvaguardia, la tutela e la rinascita dei centri storici. Ora, queste disposizioni mi consentono, cari colleghi, di offrirvi un breve spaccato di quello che è ancora oggi il tema della ricostruzione incompleta del Belice. Ad oltre quarant'anni dal sisma, la ricostruzione dei Comuni distrutti e danneggiati dal terremoto non è stata ancora completata. Le cause di questo inspiegabile ritardo sono state individuate puntualmente dalla Commissione parlamentare sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, istituita nella XII legislatura, si afferma: «Molteplici modulazioni degli impegni di spesa, spesso stornati verso altri capitoli di bilancio, ovvero andati in perenzione amministrativa a causa dei ritardi accumulati dagli organi dello Stato lo dice una Commissione parlamentare, non una commissione di amministratori locali - nell'erogazione delle somme previste ai comuni del Belice ... Oggettivo minore impegno finanziario dello Stato a favore del Belice rispetto ad altre calamità che che hanno colpito il Paese...». Ripeto, sono osservazioni di una Commissione parlamentare. La minore erogazione rispetto a quanto stanziato emerge chiaramente dalla relazione della Ragioneria generale dello Stato del 29 febbraio 1996, dove viene chiarito che per il periodo 1968-1995 le somme stanziate a favore del Belice ammontavano a 3.100 miliardi di lire, a fronte di pagamenti effettivamente disposti per 2.272 miliardi di lire, ovvero quasi il 30 per cento in meno delle somme concretamente impiegate rispetto a quelle impegnate. Anche l'insufficiente impegno finanziario dello Stato rispetto ad altre calamità emerge dall'analisi finanziaria della relazione: i 2.272 miliardi di lire erogati per il Belice,

A conferma del mancato concreto sostegno dello Stato, il documento conclusivo della Commissione bicamerale, approvato all'unanimità il 14 marzo 1996, afferma, in fine, che: «Le popolazioni interessate dal sisma del 1968 sono state vittime di insipienza e malgoverno» e che «è stata ricostruito gran parte del territorio con soli 2.200 miliardi di lire, e di ciò deve essere dato atto alle popolazioni a alle amministrazioni locali interessate». Ma lo scenario negli ultimi anni non sembra essere cambiato. Nonostante l'VIII Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 16 ottobre 2006 abbia verificato, validando il lavoro di verifica del coordinamento dei sindaci del Belice, che il fabbisogno per completare gli interventi per l'edilizia privata ammontava ancora a 430 milioni di euro e quello per l'edilizia pubblica a 133 milioni di euro e nonostante si impegnasse il Governo la finanziaria per il 2007 ha stanziato risorse per soli 100 milioni di euro in 3 anni e la finanziaria per il 2008 ha destinato 50 milioni aggiuntivi, a valere sul fondo per l'edilizia residenziale pubblica. Le risorse stanziate non solo sono state insufficienti (150 milioni, a fronte di un fabbisogno complessivo di 563 milioni), ma sono state ulteriormente ridotte da questo Governo con la manovra di luglio a soli 88 milioni di euro! E non è tutto. I 20 milioni del 2007 non sono stati ancora erogati dai Comuni ai privati e i 30 milioni del 2008 non sono stati ancora trasferiti ai Comuni: quindi le risorse o non sono state

Nonostante gli scempi del terremoto e quelli provocati dall'inadempienza dello Stato, nonostante la perdurante presenza di ruderi e rovine, la valle sembra essere risorta come territorio agricolo produttivo, intensamente coltivato a vigneti ed oliveti, attento alle colture biologiche e costellato da insediamenti agrituristici. Altri segnali positivi vengono dalla nuova generazione di amministratori locali che, come in questo caso, si è mobilitata ed affronta con coraggio e consapevolezza la gestione di un'eredità difficile, rappresentata dai nuovi insediamenti con migliaia di case vuote, da centri storici ridotti a siti archeologici, da opere d'arte arrugginite, da ettari di suoli cementificati che costituiscono le basi delle baraccopoli. Comincia finalmente ad emergere un progetto complessivo di sviluppo locale che cerca di riannodare i fili con le radici culturali delle comunità in un processo più complessivo di lotta agli sprechi e all'assistenzialismo, fondando politiche nuove sulle peculiari vocazioni della Regione. Sulla base di questa prospettiva di svolta e di ripresa, auspico che questo Governo abbia la volontà e la forza di mettere la parola fine alla storia infinita

Signor Presidente, colleghi senatori, credo che siamo in presenza di una legge che, pur sembrando di poco conto, ha invece una grossa valenza,

rappresentato dal fatto che tante leggi, che si sono accavallate nel tempo, non consentono al cittadino, e a chi vuole mettersi dentro le leggi e conoscerle con una certa facilità,

la facilità di accesso agli atti normativi vigenti nel nostro Paese sono uno dei pilastri fondamentali per la democrazia del nostro Stato. È stato necessario l'intervento del ministro Calderoli per concretizzare questo obiettivo e noi tutti della Lega Nord Padania gliene siamo grati. Siamo fortemente convinti che questo percorso intrapreso, che ha raccolto tutte quelle sensibilità che molte forze politiche in questi anni hanno espresso sull'argomento della semplificazione, sia quello giusto. Riteniamo di stare varando una riforma che è un atto dovuto ai cittadini, un importante passaggio verso una tappa e verso un modo trasparente di agire, che deve essere uno dei mezzi per avvicinare i nostri concittadini alle istituzioni e un modo per rendere più credibile anche chi, come noi, lavora in queste istituzioni. Con questa buona politica il voto della Lega Nord è favorevole. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, nell'esame di questo Atto Senato n. 1342, che reca la conversione in legge del decreto-legge sulla semplificazione normativa,

rappresentanti del Governo, cari colleghi, che pur condividendo le finalità e l'obiettivo il nostro sarà un voto di astensione.

dai nostri concittadini con molto favore perché darà un rilevante impulso alla fondamentale esigenza di semplificare il sovrabbondante, eccessivo tessuto normativo italiano, esigenza che i Governi Berlusconi hanno sempre avvertito, come pure è stata percepita dal centro sinistra. del provvedimento, esso si inquadra nella complessa azione volta alla realizzazione di una banca dati informatica pubblica gratuita contenente tutta la legislazione italiana (progetto Normattiva) che ha preso avvio con l'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Simili banche dati sono già operanti in altri Paesi europei (ad esempio, in Francia). Attualmente sono disponibili in rete solo raccolte private, in generale non complete ed accessibili solo a pagamento. Questa banca dati, una volta realizzata, oltre ad essere consultabile gratuitamente da parte dei cittadini, fornirà al legislatore strumenti per l'attività di riordino normativo. esame affida al Ministro per la semplificazione normativa qui presente il coordinamento di tutte le attività di informatizzazione e classificazione della normativa statale e regionale in corso presso le amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda la normativa regionale, il compito della convergenza presso il dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e classificazione delle normative - compito affidato al Ministro è realizzato in cooperazione con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. La costituzione di una banca dati completa sulla normativa statale e regionale vigente si è dimostrata negli anni un obiettivo molto più complesso di quanto inizialmente previsto. Le leggi in vigore, suscettibili di essere contenute in tale banca dati, ammontano a circa 60.000 e l'Istituto poligrafico dello Stato ha preventivato un costo di 200 euro per l'inserimento nella banca dati di una singola legge, compresa la sua marcatura, mentre il costo della manutenzione informatica è stato valutato ammontare a 1.800 euro annui (sempre per singola legge). Vi è quindi un incentivo anche economico a ridurre fortemente il numero delle leggi da inserire nella banca dati. Il provvedimento in esame si colloca a valle di due specifiche azioni di semplificazione normativa, entrambe attivate mediante l'articolo 14 della legge n. 246 del 28 novembre 2005. La prima azione, di natura propedeutica, è consistita nell'individuazione (affidata al Governo) da effettuarsi entro il 2007, delle disposizioni legislative statali in vigore. Tale azione, iniziata da un Governo di centrodestra, è stata completata nel dicembre 2007 dall'allora Governo di centrosinistra che ha puntualmente presentato alle Camere la relazione governativa recante la ricognizione della legislazione statale vigente: in tutto, a quella data, circa 21.000 leggi, stimando stimando che circa un quarto di esse fossero da abrogare in quanto obsolete. La seconda azione, attivata sempre con l'articolo 14 della suddetta legge, riguarda le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi. Tutte queste disposizioni saranno abrogate entro la fine di questo anno, salvo quelle per cui il Governo riterrà indispensabile la permanenza in vigore mediante l'adozione di opportuni decreti legislativi.

Si è ritenuto che per alcune migliaia di leggi anteriori al 1° gennaio 1970 fosse inutile attendere la scadenza del dicembre 2009 e che si potesse procedere fin da subito alla loro abrogazione iniziando così a fare pulizia nel complesso legislativo vigente. L'abrogazione ha riguardato circa 2.500 leggi, a cui sono state aggiunte altre 800 leggi circa emanate fra il 1970 e il 1997, per un totale di circa 3.300 leggi, analiticamente indicate. La disposizione fondamentale del provvedimento alla nostra attenzione è quella del comma 1 dell'articolo 2, che stabilisce che a decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni legislative elencate nell'Allegato 1, salvo quelle escluse dall'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005. Si tratta di tutte le disposizioni ritenute non indispensabili emanate tra il 1861 il 31 dicembre 1947, risalenti cioè al periodo antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, in tutto ben 28.889 atti normativi di rango primario. Nell'Allegato 1 questi provvedimenti da abrogare sono elencati in ordine cronologico, con indicazione della data, del numero e del titolo (talora non integrale), senza operare raggruppamenti per materia. Apprezziamo vivamente tale intervento di riduzione dello *stock* di leggi esistenti, quasi tutte di incerta o dubbia vigenza. Apprezziamo vivamente anche il coraggio del Ministro per il metodo scelto per questa decisione: è stato buttato, come si dice, "il cuore al di là dell'ostacolo". Toccherà ora alle singole amministrazioni ministeriali effettuare entro il prossimo 16 dicembre un ultimo esame di questo enorme numero di atti normativi primari,

hanno espresso nei loro pareri qualche preoccupazione in ordine all'abrogazione di alcuni dei suddetti atti normativi. Alla Camera dei deputati, ad esempio, le Commissioni giustizia, affari esteri, difesa, finanze, lavoro pubblico e privato, affari sociali e al Senato le Commissioni affari esteri, finanze e tesoro, nonché la Commissione bicamerale per le questioni regionali. Ovviamente, signor Ministro, andrà prevista a tempo debito una nuova disposizione legislativa che consenta il recupero degli atti normativi primari ritenuti meritevoli di vigenza a seguito dell'azione di ricognizione che sui 28.889 atti normativi primari abrogati con la presente legge sarà effettuata dai singoli Ministeri. In conclusione, riteniamo che il provvedimento al nostro esame, giunto all'approvazione finale nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, costituisce un grande contributo all'azione di semplificazione normativa di cui il nostro Paese ha veramente bisogno.

Prego, senatore Ceccanti. in particolar modo, in ambito elettorale, l'ultima occasione di riforma condivisa fu quella del 1995 per le regionali -, è condivisa su una piattaforma limitata, cioè quella dell'inserimento di una clausola di sbarramento, che è analoga a quella presente nelle principali democrazie e identica a quella esistente nella legislazione elettorale per la Camera dei deputati fin dal 1993.

Per cui noi, anche dopo averne discusso in Commissione affari costituzionali, invitiamo a riaffrontare subito dopo il voto, con freddezza e con calma, la vicenda. Sappiamo bene che la dimensione delle circoscrizioni non consente un buon rapporto tra eletti ed elettori; in particolar modo ci sono alcune aree sistematicamente sottorappresentate, come la Sardegna. Sappiamo che la formula elettorale è tale da provocare uno slittamento di seggi

dovranno essere affrontati con calma all'indomani del voto, valutando, anche con esperti, il rendimento del nuovo sistema elettorale, i pregi ed i limiti che esso ha denunziato. L'importante nel frattempo, visto che l'ottimo è nemico del bene, è che conduciamo in porto questa riforma condivisa.

avverto che sono da ritenersi improponibili per estraneità alla materia oggetto del provvedimento in esame emendamenti ed ordini del giorno che non abbiano a riferimento modifiche all'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, relative all'introduzione di una soglia di sbarramento per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. In particolare, sospendo la seduta. il meccanismo di accesso ai contributi elettorali, la ridefinizione delle circoscrizioni elettorali, le firme a sostegno delle candidature, la modifica del sistema delle preferenze, la modifica della legge elettorale dei due rami del Parlamento, l'introduzione di un meccanismo di alternanza delle candidature tra donne e uomini nella composizione delle liste, le minoranze linguistiche. Pertanto, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, sono improponibili i seguenti emendamenti: 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.108, 1.109, 1.110, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.200, 1.131, 1.135a, 1.221, 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102 e gli ordini del giorno G101 e G102. Colleghi, a questo punto, mancando

avremmo francamente preferito discutere qui oggi una proposta organica di riforma del sistema elettorale europeo per l'Italia. Così non è. Continuiamo a rilevare un certo strabismo nell'operato di questo Governo, che non riesce mai a presentarci progetti organici di riforma. Avrei, inoltre, auspicato un dibattito più ampio e proficuo, che ci consentisse di approfondire il ruolo che l'Italia può e deve svolgere in Europa, nell'interesse nazionale e nel più generale interesse europeo. Per quanto attiene strettamente a questo disegno di legge, va innanzitutto rilevato che, come al solito, i tempi sono strozzati, tempi che impediscono a questo Parlamento di produrre un lavoro proficuo. Questo anche per sottolineare che alzare la soglia di sbarramento è certamente opportuno per non frammentare in modo eccessivo la rappresentanza della Delegazione nazionale ed avere conseguentemente un maggior peso in Europa, è vero che non dobbiamo votare per esprimere un Governo in senso stretto, ma è anche vero che, nel corso degli ultimi trent'anni, il peso del Parlamento europeo è enormemente cresciuto e si configura oggi come un vero e proprio legislatore, unitamente al Consiglio dei ministri. In quanto tale, incide su materie che rivestono la più grande rilevanza nella vita interna di ciascun Paese. Ciò anche alla luce delle regole interne di funzionamento del Parlamento europeo: infatti, il cosiddetto metodo d'Hondt è quello in uso per attribuire secondo un criterio proporzionale le cariche ai Gruppi ed alle Delegazioni nazionali. Ciò significa che quanto più è ridotta la presenza italiana a causa della frammentazione, tanto più l'Italia diminuisce il proprio peso specifico. Siamo quindi in presenza di un sistema che avvantaggia i Gruppi più grandi, così come, all'interno dei Gruppi, avvantaggia le Delegazioni più numerose. È anche questa la ragione della maggiore influenza di altri Paesi europei, che pure hanno lo stesso numero di parlamentari eletti. Ho voluto dire ciò, in premessa, per sottolineare il nostro accordo sulla soluzione trovata alla Camera dei deputati. La valutazione positiva su tale accordo non può esimerci, però, da alcune ulteriori valutazioni. In primo luogo, sarebbe stato opportuno procedere verso una più adeguata distribuzione dei collegi elettorali, per garantire una migliore rappresentanza territoriale e quindi la vicinanza dei cittadini alle istituzioni europee; in secondo luogo, per prevedere, così come ratificato in sede europea, clausole di riequilibrio della rappresentanza di genere. Non si tratta certamente di dettagli tecnici, ma della revisione di un sistema che tenga conto dei fondamentali criteri democratici della rappresentanza: partecipazione dei cittadini, non discriminazione per le donne e le minoranze, considerazione e valorizzazione dei territori. Inoltre, credo non dovremmo dimenticare, né sottovalutare il ruolo dei Parlamenti nazionali e le procedure previste in materia di controllo dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. In tal senso, penso che dovremmo meglio organizzare il raccordo con la Delegazione nazionale al Parlamento europeo, riprendendo con più forza, dato il mutato quadro legislativo europeo, la regola degli incontri a cadenza regolare, tra i parlamentari europei e le istituzioni italiane, in particolare la pertinente Commissione di questo Senato. In questo quadro, il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali stabilisce una serie di obblighi di informazione e misure di trasparenza che dovrebbero mettere le Assemblee dei Paesi membri in grado di esercitare pienamente la propria funzione di controllo sui rispettivi Governi. Rispetto al Trattato costituzionale si è, infatti, convenuto di estendere i tempi previsti per l'esame dei progetti di atti legislativi da parte dei Parlamenti nazionali, prima che gli stessi vengano iscritti all'ordine del giorno del Consiglio nell'ambito di una procedura legislativa. Sul piano del controllo della proporzionalità e sussidiarietà, oltre al meccanismo di controllo politico *ex ante* già previsto dal Trattato costituzionale in favore dei Parlamenti degli Stati membri, il Trattato di Lisbona aggiunge un'ulteriore procedura che prevede che qualora una maggioranza semplice dei voti espressi dai Parlamenti nazionali contesti la proposta della Commissione per mancato rispetto del principio di sussidiarietà, tale proposta possa essere mantenuta, modificata o ritirata. Qualora scelga di mantenerla, la Commissione deve spiegare in un parere motivato perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. I pareri motivati dei Parlamenti nazionali e della Commissione sono sottoposti al legislatore dell'Unione che potrà bloccare la proposta con il voto della maggioranza dei voti del Parlamento europeo e del 55 per cento dei membri del Consiglio. si dovrà affrontare la frammentazione a livello dell'Esecutivo e lo scarso consolidamento del quadro istituzionale relativo alle competenze in materia europea che hanno reso più ardua l'identificazione *ex ante* e la difesa di una coerente strategia nazionale nell'arena comunitaria. Bisogna essere consapevoli che tale stile reattivo non aiuta la condivisione delle scelte europee da parte dei Parlamenti nazionali prevista nel Trattato di Lisbona ed in particolare nuoce alla trasparenza e al coinvolgimento dell'opinione pubblica. Non siamo forse i soli in Europa a dimostrare un profilo politico-amministrativo dai contorni non ben definiti, ma certo esso costituisce un *handicap* democratico non indifferente. pur non negando il nostro assenso a questa unica modifica della legge elettorale, riteniamo improcrastinabile, come da impegno assunto in Commissione affari costituzionali e come ricordato dal collega Ceccanti, ritornare sulla questione per definire compiutamente le modifiche necessarie a rendere il sistema elettorale europeo e il raccordo dell'Italia con l'Unione europea più equo, rappresentativo, partecipato e rispondente ai criteri fondamentali della democrazia in Italia e in Europa. *(Applausi

colleghi, come ho già detto in Commissione affari costituzionali ho la piena consapevolezza della solitudine, in questo caso non certo splendida, nella quale mi trovo contrastando questo provvedimento che gode di una maggioranza amplissima e la forte volontà delle forze politiche più importanti del nostro Paese del nostro Paese di portare a compimento un disegno di semplificazione dura, direi brutale della rappresentanza politica nel nostro Paese. di una volontà testarda, indisponibile ad alcuna riflessione aggiuntiva, totalmente chiusa a qualsiasi contributo emendativo è stato testimoniato non soltanto da quanto è accaduto alla Camera dei deputati qualche giorno fa, ma anche dalla stringatezza della relazione del senatore Ceccanti e dal silenzio quasi annoiato dell'altro relatore che non ha ritenuto quest'Aula meritevole di alcuna riflessione su un tema tanto delicato.

al primo giro d'orizzonte formale e sbrigativo, per quanto cortese, che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Vito, ha compiuto per verificare il grado di disponibilità delle forze politiche attorno al testo C'era tutta la possibilità di una riflessione aperta e di un'integrazione, la possibilità concreta di giungere a un testo più rispettoso delle esigenze di rappresentanza dei territori. Mi è stata però opposta in modo categorico

anche qualora ne avessero la volontà, di intervenire in questo passaggio legislativo. Tutto ciò ci è stato puntualmente confermato da quanto è accaduto alla Camera dei deputati, dove il nostro manipolo di volenterosi aveva conquistato faticosamente le firme necessarie ad ottenere il voto segreto su una serie di emendamenti

(al Senato non ci è data questa possibilità, perché i Regolamenti di questo ramo del Parlamento sono improntati a un rigore e a un'efficienza straordinaria per cui questa risorsa democratica ci è negata.). In quella sede, quando si è aperto questo spazio per tentare di inserire qualche granellino di sabbia nell'ingranaggio perfetto che avete costruito, i *leader* dei Gruppi parlamentari più importanti (e immagino anche dei partiti) sono intervenuti con una durezza senza precedenti, pretendendo dai parlamentari del PdL e del PD, firmatari di quegli emendamenti, il ritiro della firma con un atto che ne ha mortificato anche la dignità di parlamentari. *(Applausi del senatore formale e molto imbarazzante per gli stessi. Ho usato - mi è stato chiesto da un mio autorevole collega in Commissione - l'espressione «aggressività democratica» per definire questo comportamento, perché qualche volta la forza dei numeri, assolutamente rispettosa delle regole della democrazia, può essere utilizzata in modo brutale per soffocare anche quegli spazi minimi che si aprono in Parlamento all'iniziativa dei singoli parlamentari. Che tale accordo blindato faccia torto al buonsenso lo dimostra la consapevolezza che hanno i relatori del fatto che questa legge elettorale deprime la rappresentanza parlamentare delle aree meridionali, perché i meccanismi di attribuzione dei seggi, privilegiando, nel caso dell'attribuzione dei resti, il valore assoluto degli stessi e non quello percentuale, determinano costantemente lo spostamento di una quota di seggi di spettanza della circoscrizione Sud e isole, all'area del Centro e del Nord del Paese, determinando un impoverimento della rappresentanza politica di quei territori.

di premiare rappresentanti di quel territorio, come facevano i grandi partiti nazionali un tempo; così accadeva per la DC, per la quale ho militato, che garantiva sempre l'elezione ad un rappresentante della Sardegna. Oggi così non accade; ormai sono svariate volte che in Sardegna non sono eletti europarlamentari all'interno delle liste di partito. Bastava qualche piccolo accorgimento, predisporre una modifica nel sistema di computo dei resti, accettare la proposta che ho sottoscritto di separare la Sardegna dalla circoscrizione insulare per garantirle una dignitosa rappresentanza; bastava intervenire sulle circoscrizioni, riducendo queste enormi circoscrizioni e portandole a dimensione umana, regionale o al massimo di più Regioni omogenee dal punto di vista della cultura e della contiguità territoriale. Non è stato possibile. È stato possibile soltanto inserire una soglia di sbarramento durissima, quale quella del 4 per cento, che ovviamente è costruita in modo tale da penalizzare le forze minori le forze minori già assenti dal Parlamento nazionale in ragione del meccanismo di elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica e che vedono privarsi anche della possibilità di accedere ad una sorta di diritto di tribuna - perché di questo si tratta sbarramento così duro che non è assistito da una logica di efficienza dell'azione di Governo: Governo: può essere accettabile che i meccanismi di attribuzione dei seggi per il Parlamento nazionale debbano assicurare stabilità alla maggioranza e garanzia al Governo, ma il Parlamento europeo non assolve alcuna funzione come organo parlamentare che condivide la responsabilità con un Governo di chicchessia: è organo di pura rappresentanza di territori, di esperienze politiche e culturale, che ha sempre consentito consentito la partecipazione a forze minoritarie ma espressione di culture e di territori significativi.

derivato dallo sbarramento e che riguarda l'accesso ai rimborsi elettorali determina un altro *vulnus* alla democrazia del nostro Paese. Infatti, non lo condivido, non lo condivido, ma posso comprendere le ragioni politiche generali di semplificazione che hanno determinato lo sbarramento al 4 per cento: ridurre la frammentazione ed accompagnare ulteriormente questo processo bipolare che processo bipolare che incoraggi l'aggregazione attorno ai partiti più grandi; ma impedire l'accesso al finanziamento pubblico per le forze politiche che concorrono alle elezioni e che raggiungono una quota di consenso dignitosa impedisce perfino le condizioni minime della competizione, perché l'accesso al finanziamento pubblico è garanzia di trasparenza nel finanziamento dell'attività politica e di democrazia. È una legge liberticida, una legge partorita contro le minoranze, una legge che semplifica le forze politiche e semplifica la democrazia, per quanto mi riguarda riducendone la portata. Signora Presidente, in conclusione, noi abbiamo una proposta che mantenere intatti i princìpi, salvaguardando i meccanismi di rappresentanza territoriale, in linea con il processo federalista; abbiamo proposto un emendamento, che sarà presentato all'Aula e che credo possa costituire una clausola di salvaguardia per garantire che anche le esperienze legate al territorio, ove siano caratterizzate da un'autentica capacità di rappresentanza, possano avere accesso al Parlamento europeo e contribuire a costruire l'anima europea.

di opposizione a questa riforma (con rispetto parlando) della legge elettorale. Utilizzerò molto spesso la relazione (che non c'è stata riproposta quella che è stata chiamata un'integrazione era soltanto un paragrafo della relazione) con la quale è stato presentato questo disegno di legge, proprio perché ritengo che codifichi ciò che è già stato, e giustamente, denunciato dal senatore Pistorio, e cioè decisioni prese altrove sottoposte alla ratifica delle Aule parlamentari (ringrazio, ancora una volta, il senatore Pistorio per aver fatto la cronaca di quanto avvenuto alla Camera dei deputati). La conclusione della relazione cita l'articolo 49 della nostra Costituzione, dove si dice che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». La citazione di questo articolo viene a seguito di questo ragionamento, più volte ricordato, soprattutto prima che si arrivasse alla necessità di questa riforma (con rispetto parlando) della legge elettorale (riforma che era nell'aria non da Natale ma almeno dall'inizio di questa legislatura, visto e considerato che la scadenza delle elezioni per il Parlamento europeo è fissa ogni cinque anni): «Ridurre la frammentazione» - si legge nella relazione - «al di là di obiettivi di governabilità ed efficienza». La nostra legislatura passerà alla storia per essere stata la legislatura dell'efficienza, che è la peggior nemica dell'efficacia. L'altro giorno,

affinché i partiti possano svolgere quel ruolo di sintesi degli interessi (a tutti i livelli), che la Costituzione assegna loro, non solo quando c'è da scegliere un Governo, perché tale requisito rende possibile quel ruolo di cerniera fra Stato e società che i partiti sono chiamati a svolgere e riduce i micro-personalismi che spingono invece a lasciare da parte la tutela degli interessi generali».

rimarrà di un determinato ammontare, ma che, in virtù della soglia o dello sbarramento al 4 per cento, verrà ridistribuito fra i soggetti minori. Io auguro di cuore (ammesso e non concesso che si facciano queste cose, specie di martedì 17), a tutti coloro i quali insistono quotidianamente nell'affermare di essere l'unica opposizione a questo Governo, di raggiungere questo 4 per cento, perché, come si dice in alcune Regioni molto ben rappresentate nel nostro Parlamento, c'è il rischio che possiate uscire dalle tornate elettorali "cornuti e mazziati". Infatti, dopo aver denunciato questo Governo come quello peggiore e che ci vessa quotidianamente, cari colleghi dell'Italia dei Valori, avete acconsentito a che si arrivasse a questo

con il quale vi siete messi d'accordo per cambiare la legge - che è il peggiore possibile, e contro il quale solo voi, cancellando i Radicali (come forse stava cercando di fare anche il senatore Pistorio), siete l'unica opposizione. Complimenti! Sarebbe bene che questi dibattiti avvenissero a reti unificate, proprio perché così si saprebbe

Si dice - e lo ha ripetuto poco fa il senatore Ceccanti - che raramente si era arrivati a conclusioni condivise relativamente a modifiche delle legge elettorali.

con tempi ristretti rispetto alla corretta operatività, che in astratto sarebbero da evitare, ma che talora in concreto appaiono preferibili, purché vi sia largo consenso, ad uno *status quo* negativo»; ed infatti il largo consenso lo avete tranquillamente trovato. Ciò che non si desume da questa relazione è quale sia la necessità e l'urgenza, a tre mesi - anzi, a due mesi e mezzo - dalla chiusura delle liste per il Parlamento europeo, di apportare tutte queste modifiche. Ebbene, già che c'eravate, considerato che la stragrande maggioranza dei colleghi qui presenti, e di quelli della Camera, era d'accordo, non si capisce perché non sia stato possibile ridisegnare i collegi. 72-73 collegi sareste riusciti ad andare contro quei partiti politici che voi ritenete essere quelli dell'articolo 49 della Costituzione, ma che invece sono quelli della consociazione e della spartizione quotidiana

Avviandomi a concludere, signora Presidente, il tempo a disposizione per fare queste modifiche non è sembrato opportuno per apportare altri tipi di cambiamenti, che sarebbero stati quelli per legare - e questo sarebbe stato l'unico modo di mandare finalmente degli europarlamentari dalla Sardegna

provvedimento, e spero che la coscienza di molti, appartenenti tanto alla maggioranza quanto all'opposizione, si svegli al momento del voto (non tanto sugli emendamenti che poco cambiano, ma sul provvedimento nel

dell'Europa delle Nazioni e del Partito popolare europeo appartenete, volete o vorreste appartenere in futuro. Quindi, tutta l'argomentazione relativa alla possibilità di rappresentare meglio gli interessi del nostro Paese a Bruxelles o a Strasburgo, la potete mettere da parte. Ciò certifica ancora una volta il ratto: non soltanto avete portato via soldi, ma porterete via diritti civili e politici

della legge elettorale per le politiche nazionali, a essere classificato comunque come 4 per cento, perché la folla, convocata dalla RAI e da Mediaset, lo invoca. Di certo sarà utile, quando vorrete degnarci di riprendere in mano la riforma (con rispetto parlando), valutare sotto tutti i punti di vista - primo fra tutti quello della Costituzione - il rendimento di questa pessima riforma di legge elettorale.

ha detto anche il senatore Pistorio, con particolare riferimento alla formula elettorale, al «ritaglio» delle circoscrizioni e all'espressione del numero di preferenze sino a tre, che avvantaggiano le Regioni e le zone all'interno di esse più popolose a discapito di quelle meno abitate.

sul rimborso delle spese delle forze politiche che non raggiungono il 4 per cento sia stato per ora accantonato. Spero che possa in seguito diventare intervento fattivo. Quindi, c'è un ulteriore problema che contrasta la possibilità materiale di far valere le proprie idee e di concorrere anche se non si raggiunge il 4 per cento (ritengo che anche questa sia un'opinione abbastanza personale).

Non soltanto perché la soglia del 4 per cento ed oltre, come soglia implicita, è presente in tutti i grandi Paesi europei (mentre i Paesi più piccoli hanno apparentemente soglie minori perché eleggono

importante raggruppare, mettere una soglia, fortificare la rappresentanza politica dei parlamentari italiani al Parlamento europeo? Perché il Parlamento europeo, diversamente da quanto si pensi, è un'istituzione cruciale nella politica comunitaria e lo è divenuto sempre di più; esattamente al contrario di quanto si pensi, il Parlamento europeo ha poteri di codecisione, insieme al Consiglio dei ministri, per importanti politiche pubbliche (ad esempio, per il finanziamento del mercato comune), e gli esiti di queste codecisioni e di questa dimensione di Governo sono la legislazione europea attuale che determina, così potentemente e in grande misura, la legislazione dei singoli Stati. Quindi, la prima obiezione dei molti che, anche in questa sede, dicono no alla soglia, perché un Parlamento che rappresenta è sufficiente, è un'obiezione storicamente storicamente e contingentemente infondata e, permettetemi di dirlo, maggiormente infondata oggi in questa crisi così pesante e a causa della quale le istituzioni comunitarie dovranno essere Quindi, diventa essenziale avere, all'interno dei principali partiti parlamentari europei (perché sono partiti parlamentari), influenti rappresentanze nazionali. o i parlamentari italiani fanno massa critica dentro i partiti parlamentari europei oppure l'inevitabile marginalità decisionale dei partiti italiani, come è ora e come è stata negli ultimi decenni in Italia, sarà ancora più evidente.

far massa critica e rendere incisiva la rappresentanza del suo Parlamento nazionale. È poi importante avere - questo non lo dice la legge, lo dico io - una classe di parlamentari

selezionare solo per censo le forze politiche. Posso non raggiungere la soglia del 4 per cento ma devo, ciò nondimeno, sapere di poter avere le risorse per concorrere, per presentare i miei candidati, le mie idee, i miei progetti. Questo è un punto da

e guai a noi se pensassimo sensato polverizzare la rappresentanza italiana, oggi che siamo nel cuore di una crisi economica e politica di inaudita grandezza.

che introduce la soglia di sbarramento al 4 per cento, consentirà innanzitutto di allineare il nostro sistema di voto a quello di molti Paesi europei. Ma, accanto a questo, c'è un altro obiettivo da centrare: mi riferisco all'evoluzione del sistema politico del nostro Paese, che da questa riforma potrà trarre la spinta necessaria per strutturarsi e finalmente compiersi. Ai partiti, che animati dalla preoccupazione legittima di difendere l'identità, collegano alla nuova norma sullo sbarramento il rischio di essere estromessi dalla rappresentanza europea, vorrei ricordare che l'identità non è in questione perché essa resta sempre ben impressa nel codice genetico di ciascuno di noi e di ciascuna forza politica.

Resto convinto che la nuova norma sullo sbarramento in campo politico debba stimolare una spinta all'aggregazione piuttosto che alla divisione, in modo da favorire un sistema bipolare compiuto, strutturato su due blocchi politici di centrosinistra e centrodestra chiaramente distinguibili sulla base di proposte politiche definite ed alternative; nella consapevolezza che, esaurita la stagione dei partiti a forte connotazione ideologica, ora è il programma, l'identità, il progetto l'elemento cardine per imbastire e qualificare le alleanze politiche. A mio avviso, è pienamente compiuta, anche se non sostenuta - avverto una certa distrazione sul piano politico-culturale - con eguale convinzione dalle forze politiche, quella che Aldo Moro definì "la terza fase", che segna l'avvio della democrazia dell'alternanza, con la possibile articolazione di due coalizioni contrapposte che hanno a cuore gli interessi generali del Paese e non i propri

Per farlo occorre una semplificazione del sistema politico e la riforma per le elezioni europee può essere utile ad innestare la marcia giusta per arrivare a definire, sulla strada delle riforme da attuare, una nuova legge elettorale a livello

la questione vera da affrontare, una domanda che si leva dalla società ma che non trova risposta nell'attuale legge elettorale nazionale, che prevede liste bloccate formate da cooptati e che, dunque, creano dannose rendite di posizione. un sistema che ha contribuito e contribuisce ad acuire la perdita di credibilità della politica e ad aumentare la distanza tra elettori ed eletti,

obbliga ad una riflessione che non sia solo una mera presa d'atto, ma si traduca in una spinta a fare, ad intervenire per cominciare ad invertire la rotta, soprattutto in riferimento alla frammentarietà del quadro politico, alla quale, proprio focalizzando l'attenzione sulla necessità di recuperare il rapporto tra elettori ed eletti, tra eletti e territorio, vanno posti degli argini. restituendo alla politica il compito, il valore di farsi interprete delle istanze della collettività e non di gruppi di potere, e ai partiti il loro ruolo definito mirabilmente dalla nostra Carta costituzionale nell'articolo 49, ma stando bene attenti a non disperdere le energie in mille rivoli, in partiti e partitini che circoscrivano la loro esistenza alla difesa di piccole sigle battere Berlusconi è importante, ma la priorità oggi, anche per uscire dalla balcanizzazione del quadro politico, è la difesa di principi fondamentali della democrazia che vengono minacciati ogni giorno. che, facendo leva sui valori fondanti, sulla storia culturale e politica del Paese, può costruirsi un blocco politico alternativo a quello di destra sovente populista e, mi sia consentito, ancor più spesso irresponsabile rispetto alla salvaguardia della della democrazia e degli equilibri istituzionali previsti dalla Costituzione. In questo senso la crisi può, anzi deve, servirci come opportunità per operare il ripensamento di un sistema che, a mio

il motivo per cui il mio voto sarà favorevole - deve rappresentare la prima tappa di un viaggio impegnativo, ma senza dubbio affascinante. Colgo infine l'occasione,

siamo di fronte ad una pseudo riforma della legge elettorale europea poiché il termine riforma, nella sua autentica accezione, avrebbe significato mettere mano con coscienza e consapevolezza ad un sistema elettorale delicato e complesso, qual è quello che riguarda appunto le elezioni per il Parlamento europeo, tenendo presenti alcune delle questioni che da tempo non sono state risolte dai nostri legislatori nazionali. Ma, guarda caso, in questo momento è stato molto più produttivo e naturalmente più efficace, per certe finalità e per certi scopi, arrivare ad una modifica della legge elettorale introducendo semplicemente, *sic et simpliciter,* una soglia di sbarramento al Come ci siamo arrivati, signora Presidente? Ci siamo arrivati per la volontà di due *leader,* uno di centro destra e uno di centro sinistra, che hanno fatto un accordo che non ha assolutamente preso in considerazione la volontà non solo delle forze presenti in questo Parlamento, ma anche e soprattutto di quelle che in questo Parlamento non sono potute entrare per una legge elettorale, fatta anche quella a colpi di mano, all'ultimo momento, che ha visto scomparire dal Parlamento la Sinistra radicale, i Verdi e altri. Noi Repubblicani europei, come i Radicali, siamo presenti all'interno del Partito Democratico, ma non siamo Partito Democratico: siamo forze alleate del Partito Democratico e su questo punto non siamo stati consultati, così come non lo sono stati i cittadini italiani. Ci troviamo una soglia di sbarramento al quattro per cento, si dice, perché è necessario lottare contro la frantumazione delle forze politiche e si confonde pluralismo con frantumazione. Pluralismo non è frantumazione secondo quanto recita la nostra Costituzione repubblicana. Voglio ricordare che i pilastri essenziali della nostra Costituzione liberaldemocratica sono contenuti innanzitutto nelle a tutti, e dico a tutti, il diritto di esprimere le proprie opinioni e di confrontarsi; è riconosciuta a tutti, e dico a tutti, la garanzia di poter esercitare i diritti di libertà

Per forze che appartengono alla mia tradizione, quella democratica repubblicana (come - penso - a quella dei radicali), per forze che sono libertarie e hanno questo concetto di libertà nel loro DNA (libertà repubblicana, intendo naturalmente), è assolutamente impossibile aderire a progetti che significano *reductio ad unum* a destra o a sinistra dentro il partito maggioritario, rinunciando alla propria identità, alla propria vocazione, ai propri princìpi, ai propri valori di riferimento. Io credo che nel nostro Paese la libertà per tutti e per ciascuno di poter esprimere i valori, i propri convincimenti, i propri convincimenti, posizioni non partitocratiche, ma culturali, perché afferenti a dei valori democratici, debba essere assolutamente garantita. Questo è un colpo di mano, naturalmente per fini molto poco nobili, che non sono né la governabilità (perché non c'è un Governo da sostenere in Europa), ma sono semplicemente la possibilità di lucrare alle spalle dei cosiddetti piccoli, dei cosiddetti frammenti, dello "zero virgola" (come qualcuno diceva). Io sono ben orgogliosa di essere uno "zero virgola" e intendo restare uno "zero virgola" in questo Paese se significa essere persona libera. La possibilità di esprimere un pensiero divergente noi la dobbiamo difendere, perché questa è lotta contro l'assuefazione, contro l'omologazione, contro il qualunquismo becero anticulturale e antidemocratico che ha ridotto questo Paese in ginocchio. In Italia, signora Presidente, Presidente, c'è un avviamento costante e progressivo verso una deriva che noi abbiamo definito più volte populista e peronista, sotto la spinta di forze che sono nichiliste e quantomeno qualunquiste che, qualunquiste che, sotto l'egida di un vergognoso incontro o matrimonio (se lo vogliamo definire in termini più prosaici) tra il trono e l'altare, stanno trascinando il Paese fuori dal contesto di quegli Stati liberi tra l'indifferenza generale. Contro questa indifferenza, che si basa soprattutto e fonda il suo successo sull'ignoranza, sull'incultura, dobbiamo continuare a lottare. Nel nostro Paese c'è peraltro un intreccio che tutti denunciano ma poi quando fa comodo mettiamo in disparte; un intreccio vergognoso tra la politica e i *mass media*, per cui tutti coloro che saranno esclusi grazie a questo quattro per cento non avranno più voce, non avranno più alcuna possibilità di partecipare ad una trasmissione televisiva, di avere una riga su un giornale, non avranno quindi possibilità di esprimere quelle opinioni che la Costituzione garantisce a tutti ed a ciascuno. il silenzio dovuto al fatto che uno si tappa la bocca o c'è il silenzio dovuto al fatto che qualcuno te la "tappa"; in questo caso c'è l'hanno "tappata" o vogliono "tapparcela". Nel nostro Parlamento ci sono forze che hanno dietro le loro spalle una storia fatta di valori, che non sono frutto di un retaggio economico, né possono essere ascritte a partiti azienda o a partiti francobollo che nascono all'ultimo minuto, perché ci sono battaglie battaglie storiche che stanno alle nostre spalle fatte della condivisione di valori democratici e repubblicani ai quali non possiamo naturalmente non fare più riferimento. Noi vogliamo continuare ad essere noi stessi, vogliamo partecipare con le nostre forze, con le nostre idee. Se poi la legge non ce lo consente perché non raggiungiamo un *quorum*, va bene; ma, cara Presidente, per eleggere un parlamentare europeo la soglia di sbarramento è già stata fatta, perché i seggi sono stati portati a 72 e per eleggere un Parlamento europeo ci vogliono 370.000-380.000

di un progetto per l'Europa, di un'idea di Europa che per noi deve essere l'Europa dei popoli e l'Europa naturalmente fondata su un concetto di federalismo che è ben diverso da quello che si sta introducendo nel nostro Paese. Vogliamo un'Europa che sia in grado di tenere la testa alta, di competere a livello mondiale in termini politici, perché compete come continente. Questa è l'Europa che vogliamo come Repubblicani Europei. È la stessa Europa che vuole il Partito Democratico? È la stessa Europa che vuole il partito di Berlusconi? Non lo so. Voglio poter dire la mia e voglio che il popolo italiano ascolti anche una voce divergente.

Signora Presidente, credo che stasera non possa sfuggire alla nostra Assemblea che stiamo discutendo della credibilità istituzionale del Parlamento europeo, un consesso che non sempre è stato eletto dal popolo, visto che nel suo esercizio originario veniva nominato dai Parlamenti nazionali. Credo nel Parlamento europeo eletto dal popolo e nella sua credibilità. Sono conscio, però, come molti di noi, che questa credibilità il Parlamento europeo la stia lentamente perdendo anche per le modalità della sua elezione con suffragio universale. È difficile la rendicontazione politica del parlamentare europeo; è difficile la sua elezione; è difficile il rapporto con il collegio; a volte, una identificazione degli interessi legittimi che porta. Avevo presentato, insieme ad altri colleghi, un emendamento - poi ritenuto inammissibile che, proprio in funzione di ridare credibilità all'espressione nazionale del Parlamento europeo, mirava a tirare fuori dalla circoscrizione insulare l'isola di Sardegna. La chiamo così perché lo stato particolare di isola è riconosciuto dal Trattato di Amsterdam, perché la Sardegna è un'isola vera, circondata dal mare, molto distante dal continente italiano e dal resto dell'Europa e, a differenza di altri territori insulari, come la Sicilia, per la sua collocazione dentro un'infelice *constituency* elettorale, normalmente non riesce ad esprimere parlamentari europei.

L'isola di Malta, che ha 395.000 abitanti, esprime di diritto cinque parlamentari europei. Io mi rammarico per la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento, che non consente di portare alla delibera del Senato la nostra questione. Concludendo, le dico, Presidente, consapevole che le decisioni della Presidenza sono inappellabili su questo punto, che quel modo restrittivo di applicare l'articolo 97 del nostro Regolamento rende praticamente vana questa discussione. Alla Camera hanno discusso per poi concentrare la decisione su nove disegni di legge. Noi non possiamo applicare il nostro Regolamento fingendo e - mi consenta di dire - simulando che siamo impossibilitati a discutere su nient'altro che l'articolo 21 di una legge di trent'anni fa. Non è questo il modo di legiferare, assumendoci pienamente le nostre responsabilità. a parlare il senatore Vita. di un argomento molto delicato (riguarda le libertà di espressione), che non è una mera pratica burocratica. Certo, capisco, accordi politici più generali hanno influenzato eccome questa materia, però è bene che io sottolinei qui con molta amarezza il fatto che forse questo argomento avrebbe meritato ben altro approfondimento e, soprattutto, ben altro tempo. Il tempo è una variabile sempre essenziale nella politica, così come nelle cose della vita. Questo stesso tema, qualche mese fa, avrebbe avuto un sapore assai diverso; ora, così ravvicinato è il termine della scadenza elettorale cui fa riferimento il disegno di legge atto Senato n. 1360, che ogni iniziativa

questa volta è bene sottolinearlo - persino dai soggetti o dagli oggetti della ipotetica tutela

andare a riflettere, come ha detto anche la senatrice Sbarbati, sulla opportunità, sulla natura, sulla soggettività di questa o quell'altra forza esclusa dalle Assemblee parlamentari: certo è che, all'ultimo, è difficile supporre che vi possa essere una consapevolezza adeguata del rischio che la nostra stessa struttura democratica corre. Tra l'altro, in una estemporaneità della nostra normativa elettorale, fosse questo un

il nostro Paese, sotto il profilo anche elettorale. Due emendamenti, signora Presidente, colleghe e colleghi, sono stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza

ovvero il finanziamento per chi, concorrendo anche senza raggiungere il quoziente, arriva almeno alla soglia non così banale del 2 per cento. Formulo quindi una protesta: non voterò, Presidente, colleghe e colleghi, questo provvedimento, perché mi pare profondamente sbagliato per il suo tempo e anche per quello che dice. Come ho detto, qualche mese fa, avrei voluto partecipare ad una discussione assai diversa, oggi mi sento in dovere di fare questo richiamo, che non è solo un richiamo di coscienza: è un richiamo rispetto ad una regola democratica, e cioè il fatto che vanno rispettate le diverse forze in campo e va permesso che anche chi non ha raggiunto in elezioni recenti la soglia per entrare nelle Assemblee nazionali possa,

e anche una protesta: è un modo di riflettere su temi così delicati quanto meno incerto, non degno, insomma, dalla grande tradizione che le nostre Assemblee hanno, anche sotto il profilo della regolazione della nostra vita elettorale.

le elezioni europee di giugno 2009

un momento di grandiosa celebrazione della democrazia. 495 milioni di cittadini e cittadine saranno chiamati ad eleggere i propri rappresentanti e 27 Paesi saranno interessati alla consultazione. Sono le prime elezioni a cui Romania e Bulgaria partecipano insieme agli altri Stati membri e 736 eurodeputati verranno eletti. momento elettorale che per i numeri risulta secondo, nel panorama delle democrazie compiute, soltanto all'India. L'imponenza dei numeri, tuttavia, non può servire da schermo alle problematiche che ancora rimangono vive in questa tornata elettorale, la quale si svolge a distanza di trent'anni dal primo suffragio elettorale diretto del 1979. Mi riferisco, tra le altre, all'assenza dei veri partiti paneuropei, al calo della partecipazione elettorale, alla difformità dei sistemi elettorali tra i vari Paesi membri, nonché alla sensazione diffusa che, nonostante si vada ad eleggere la più grande Assemblea paneuropea, la competizione rimanga ancorata a strette logiche nazionali. È in tale ottica, cari colleghi, che mi appresto a discutere il disegno di legge n. 1360, privilegiando gli aspetti europei del disegno di legge stesso e posponendo ad un secondo momento la discussione sui rilievi nazionali dei quali comunque riconosco l'importanza. Inizio con una considerazione amara: negli ultimi sedici anni l'affluenza alle urne europee è a dir poco precipitata, ma nessuno se ne accorge o se ne vuole accorgere: dal 63 per cento del 1979 arriviamo fino al 45, 6 per cento Perché questo disincantamento dell'elettorato? Perché questa disaffezione del cittadino europeo verso un evento che, come dicevo, potrebbe rappresentare il massimo fulgore del più importante processo democratico sorto dalle ceneri di un conflitto e arrivato ad una comunione di finalità, principi e meccanismi istituzionali? Parte della ragione consiste certamente nella debolezza della comunicazione, visto che di Europa e di Parlamento europeo si parla poco e, purtroppo, male. L'altra causa risiede nell'architettura costituzionale dell'Europa, caratterizzata da deficit di democrazia. Oggi, infatti, il Parlamento non ha poteri forti e non esprime un Governo, in quanto la Commissione viene formata su designazione dei Governi nazionali e il Consiglio è diretta appendice degli stessi. infine, influito la frammentazione delle campagne elettorali, la differenziazione delle procedure elettorali e l'assenza di liste comuni su tutto il territorio comunitario. Mi chiedo allora come potrà la modifica che il disegno di legge n. 1360 apporta alla nostra legge elettorale cambiare questo quadro. Cosa si dovrebbe fare in futuro per costruire non l'Europa dei vertici, delle burocrazie, degli interessi nazionali, ma l'Europa dei popoli che crede fermamente nella possibilità per i Paesi europei di unirsi e svolgere una crescente funzione nel quadro della comunità mondiale? La prima necessità sarebbe quella di arrivare ad una procedura elettorale uniforme per l'elezione del Parlamento europeo. L'articolo 138 del Trattato CE ha conferito all'assise il potere di elaborare un progetto di procedura elettorale uniforme, ma i vari tentativi si sono inesorabilmente scontrati con il Consiglio dei ministri e, in particolare, con il suo paralizzante voto all'unanimità. momento, pertanto, si è proceduto ad un semplice ravvicinamento dei sistemi nazionali sulla base di principi comuni quali elezione a scrutinio di lista, uninominale preferenziale, carattere proporzionale del voto, possibilità di prevedere una soglia minima per l'attribuzione dei seggi non superiore al 5 per cento. Con il disegno di legge n. 1360 si è mantenuto un sistema di tipo proporzionale, si è lasciato impregiudicato il sistema delle preferenze, la cui modifica ci ha visti nella discussione alla Camera risolutamente contrari, ed é stata introdotta la soglia di sbarramento al 4 per cento. Questa soglia avvicina l'Italia alla maggioranza degli altri Paesi membri; avremmo preferito una soglia più dolce, ma nel merito della misura siamo d'accordo, in quanto ha un effetto di aggregazione partitica, semplificazione del quadro dei Gruppi parlamentari e riduzione di micropersonalismi. Tale parere positivo va letto anche in un'ottica più generale; questa non può essere considerata un'operazione limitata a indicare esclusivamente determinati meccanismi e procedure legate all'espressione tecnica del voto, né può prescindere dalla natura e dalla finalità del sistema politico e del processo di integrazione comunitaria. È evidente, cari colleghi, che esiste una relazione intima tra l'esigenza dell'elezione diretta dell'assise con procedura uniforme e una maggiore attribuzione di competenze al Parlamento europeo. Con il Trattato di Lisbona, la cui entrata in vigore ci si auspica possa avvenire nel 2009, il Parlamento europeo vedrà rafforzata il suo ruolo di colegislatore. Ad esso si aggiungeranno due funzioni politiche cruciali: il Presidente della Commissione dovrà essere designato tenendo conto del risultato delle elezioni europee e il potere costituente sarà esercitato anche dall'Assemblea, oltre che dai Governi e dalla Commissione europea. All'interno delle famiglie politiche europee (popolari, socialisti, liberal-democratici, verdi, comunisti) la capacità di influenza dei Partiti nazionali è poi legata alla loro coesione politica e la frammentazione è inversamente proporzionale all'esercizio di questa influenza. Inoltre, al centro di ogni democrazia rappresentativa si colloca il potere del popolo di scegliere, attraverso l'esercizio del voto, il Governo e tale potere si esercita, non solo in entrata, ma anche in uscita. Una maggiore razionalizzazione delle forze politiche in Parlamento e l'aver legato la nomina del Presidente della Commissione al risultato delle elezioni europee permettono di ottenere quella che in inglese si chiama *political accountability*. In vista del voto che avrà luogo nel giugno del 2009 sarebbe importante che coalizioni di partiti europei proponessero agli elettori i loro candidati alla Presidenza della Commissione, associando a questa proposta quella di un programma per la legislatura, in modo da permettere agli elettori di esprimere con consapevolezza la loro scelta e al nuovo Presidente di rispondere nella sua opera ai cittadini che lo hanno indirettamente

(quella della soglia di sbarramento) e che toccano maggiormente tematiche di interesse nazionale. Con il disegno di legge n. 1360 si è normato esclusivamente sull'introduzione della ma si sono lasciate impregiudicate le altre parti della legge n. 18 del 1979, poi novellata dalla legge 27 marzo 2004, n. 78: la definizione delle circoscrizioni elettorali, le modalità di presentazione delle candidature, la presenza di candidature femminili nelle liste, nonché la tutela di liste rappresentative di minoranze (il rapporto tra le stesse potrebbe sotto alcuni aspetti rivelarsi problematico). Già sul primo punto - quello relativo alle circoscrizioni elettorali - si rileva come la divisione delle stesse in cinque maxiaree non consenta un rapporto fiduciario stretto tra elettori ed eletti e neghi quindi quella *accountability* di cui si diceva sopra. In particolare - mi rivolgo anche alle preoccupazioni espresse dai colleghi - si potrebbe citare, come già hanno

Diceva bene il collega Vita: noi abbiamo lavorato di fretta, come sempre con questo Governo.

Nella nostra legislazione tale principio è ripreso, ma, come solitamente avviene per le questioni di genere, soltanto in linea teorica. In conclusione, rimangono ancora dei punti controversi su cui, a seguito di questa prima parziale riforma della legge elettorale, le nostre Camere potrebbero e dovrebbero tornare a discutere in futuro, perché la rappresentanza politica costituisce l'elemento chiave del futuro di un'effettiva comunità dei popoli e

noi siamo chiamati a razionalizzare la rappresentanza dei cittadini, come è nello spirito delle modifiche apportate alla legge n. 18 del 1979. Una forza popolare per eccellenza, qual è la Lega Nord, non può esimersi dal soppesare con un'attenzione del tutto particolare (direi con autentico scrupolo democratico) la portata di questo cambiamento. Nel considerare le correzioni al vigente sistema elettorale delle consultazioni europee, neppure per un attimo abbiamo inteso sottovalutare, tanto meno sottacere, l'effetto di ridimensionamento della rappresentanza partitica già implicito nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. Al contrario, come movimento di popolo abbiamo affrontato la questione di democrazia posta dalla soglia di sbarramento fissata al 4 La risposta è che questa apparente limitazione dell'espressione democratica costituisce invece, a differenza di quanto hanno sostenuto i colleghi che mi hanno preceduto, un modo superiore di adempiere alla più larga e manifesta volontà popolare. L'archiviazione dell'eccessiva frammentazione politica, con i costi e guasti che quest'ultima produce, è infatti una delle istanze più diffuse tra la popolazione, come ampiamente ribadito da tutti gli osservatori della cosa pubblica e come confermato da unanimi sondaggi, che concordano nell'attribuire un consenso semplicemente plebiscitario all'introduzione della soglia di sbarramento. Si tratta di una diga che peraltro detta le regole del pluralismo nei maggiori Paesi europei.

mentre in altri Paesi, come la Gran Bretagna, i meccanismi del sistema elettorale stabiliscono una soglia effettiva che gli esperti quantificano intorno al 10 Nella vita parlamentare delle suddette Nazioni non avrebbero diritto di cittadinanza tutti i cosiddetti partitini, i cui rappresentanti in questi giorni hanno manifestato davanti ai palazzi romani della politica, gridando alla congiura e al complotto consumato ai loro danni. Alcuni tra questi - penso a certi esponenti di Rifondazione Comunista in tempi di maggiore seguito elettorale avevano dato il proprio assenso all'introduzione della soglia di sbarramento, magari nella speranza di estromettere dalle Aule parlamentari proprio il nostro movimento. Non è andata così, Non è andata così, ma non è certo della sconfitta e dell'emarginazione altrui che ci rallegriamo. Oggi, piuttosto, abbiamo la possibilità di esprimere la nostra soddisfazione per una vittoria dei cittadini sul Palazzo. Da mezzo secolo, infatti, un popolo assisteva impotente e attonito a quelle che venivano definite alchimie delle segreterie di partito. Il cittadino che, esaurite le lusinghe della campagna elettorale, riacquista puntualmente i panni del vessato contribuente, ha sempre pagato i costi di certe scandalose rappresentazioni del malinteso pluralismo politico. Il confronto fra partiti, così sovente scaduto a guerra per bande, ha troppo a lungo visto i più piccoli fare la voce grossa tenendo in ostaggio il Governo. invece, distolto dalle sue priorità, per troppo tempo è stato impegnato in estenuanti bracci di ferro con chi ogni giorno accampava nuove pretese per sé e per le proprie clientele - come si suol dire - da Prima Repubblica. Ma il tanto atteso avvento della Seconda, più volte evocato in maniera ingannevole, solo ora comincia a manifestarsi seriamente con i segni di un cambiamento, che troverà nell'attuazione della riforma federalista il suo pieno compimento. Concludo, signor Presidente, evidenziando che, in questo senso, anche l'archiviazione del partitismo selvaggio, dei ricatti e del malcostume che gli sono propri vuole indicare come sia stato concretamente intrapreso quel cammino di rinnovamento che tante generazioni di padani e di italiani avevano appena potuto sognare.

ma dobbiamo occuparci di legge elettorale, visto che, mentre ci accingiamo a modificarla, l'Europa continua a morire nel silenzio di tutti, inclusi coloro che l'hanno sempre solennemente sostenuta; ci stiamo accostando, però, a questo tema - va detto - con idee e sensibilità che attengono più alla politica nazionale che non ad una politica europea. Sappiamo che, con la complicità della stampa, che praticamente ignora le vicende politiche europee, i nostri partiti non aiutano i cittadini italiani a seguire o a leggere la politica europea. Quando si vota per il Parlamento europeo - ce lo dobbiamo dire con molta serenità ed onestà - i cittadini si accostano al voto con valutazioni e giudizi che attengono alla politica nazionale. Bisogna ammettere che questa legge è stata dettata da logiche di politica nazionale. È vero, non non c'è dubbio; è così perché è questo il modo in cui viviamo la politica europea. Tuttora i *leader* dei partiti dicono: alle europee vedremo il risultato e quel che accadrà nel nostro partito e, nella politica italiana.

Votiamo in massa per l'Europa, ma la politica europea non ha diritto di cittadinanza nell'opinione pubblica italiana. Naturalmente è vero che la legge europea permette - e non impone - uno sbarramento fino al 5 È stato introdotto uno sbarramento del 4 per cento perché è oggettiva la necessità di semplificare la politica italiana. Nella scorsa competizione elettorale nazionale, i partiti della sinistra antagonista non hanno raggiunto il 4 per cento. Però, vorrei far notare che vi erano altri due partiti della sinistra antagonista che insieme hanno ottenuto su un consenso dell'1, 3 per cento. L'uno ha ottenuto lo 0,7 e l'altro lo 0,6. Se ci fosse stata unità, lo sbarramento del 4 per cento sarebbe stato superato. Dunque, possiamo continuare ad avere tre, quattro partiti che addirittura hanno lo stesso nome? Possiamo continuare ad alimentare personalismi che all'estero e guardati dall'estero fanno soltanto ridere? Ecco la ragione per cui sono favorevole a questa legge. Comprendo che l'*iter* che ha portato all'approvazione poteva essere più coinvolgente, più condiviso.

Mi meraviglio che qualcuno che ha tuonato contro di essa ha poi firmato il *referendum* sulla legge elettorale italiana proposta dal senatore Ceccanti. È vero che non era facile ridisegnare le circoscrizioni rendendole più piccole, ma si poteva risolvere il problema della Sardegna, ad esempio, prevedendo la preferenza unica. unica. Se anziché con tre preferenze si votasse con la preferenza unica, sarebbe stato già un modo per garantire le piccole Regioni che si trovano in circoscrizioni più ampie, come la Sardegna.

che ci accingiamo a vivere nell'*iter* di approvazione della legge sulle autonomie e, speriamo, anche in quelle che si preannunziano come modifiche costituzionali. Mi sia consentita, però,

nonostante non siano proponibili proposte, emendamenti ed ordini del giorno che attengono alla legge elettorale italiana,

che, fra le altre cose, chiedono di introdurre le preferenze o comunque di introdurre una possibilità di scelta dei rappresentanti parlamentari Ora, se non sono ammissibili emendamenti ed ordini del giorno, la parola può ancora rimanere libera. Colgo quindi l'occasione per dire a quest'Aula che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani chiedono una legge elettorale diversa con cui possano eleggere i propri rappresentanti. si determina una ferita gravissima, non solo alla democrazia del nostro Paese, ma allo spirito della Costituzione, perché la centralità del Parlamento, nel momento in cui lo stesso è nominato da tre o quattro personaggi, sia pure autorevoli, cessa di essere tale.

sulla scarsa autonomia del Parlamento che, quando è nominato, finisce per essere esclusivamente fedele, non ai cittadini, non ai territori, ma soltanto alle figure che hanno indicato i parlamentari. Non voglio fare come Catone che cominciava tutti i suoi discorsi con *delenda* *Cartago*, ma occorre che qualcuno di noi, come ha fatto il senatore Perduca per altre questioni, ricordi all'inizio di ogni seduta che questa è una ferita che va sanata.

su un tema che a me, come ad altre colleghe presenti in questa Aula, sta particolarmente a cuore: quello della rappresentanza femminile. Le elezioni europee del prossimo giugno si terranno anzitutto sulla base del Trattato di Nizza, che ha ridotto il numero di deputati europei da 785 a 736; ciò comporta alcuni adattamenti automatici da parte dei Paesi membri, non ultima la necessità di ridurre la frammentazione della rappresentanza, indirizzando i partiti politici a dar vita a Gruppi parlamentari più coesi e rappresentativi. Attualmente l'Italia è rappresentata da 18 delegazioni parlamentari,

è stato necessario per consentire un adeguamento dell'Italia agli altri Stati membri dell'Unione. Gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale la soglia di voti necessaria per ottenere un seggio, non oltre il 5 per cento dei suffragi espressi; undici Stati già praticano questa soglia, anche In altri termini, la tendenza ormai consolidata è quella di garantire una rappresentanza chiara e netta, senza indulgere a quella frammentazione politica e parlamentare, che in Italia per molti anni ha condizionato il nostro sistema democratico. Ciò che conta è la capacità di riformare e cambiare, stabilendo una prospettiva di progresso e di evoluzione politica, non solo nell'ambito nazionale, ma anche e soprattutto europeo. A questo si aggiunge la crisi economica che colpisce che colpisce indiscriminatamente i singoli partiti e interi continenti, e che sta a dimostrare che, in piena globalizzazione, occorre fronteggiare uniti gli effetti devastanti della crisi finanziaria. Il Parlamento europeo, pertanto, è chiamato a svolgere una funzione legislativa ed un ruolo di crescente importanza in una logica innovativa della rappresentanza popolare. Il semplice meccanismo elettorale dello sbarramento imprime una spinta all'aggregazione del consenso politico su un fronte dello schieramento o sull'altro, cioè quello opposto. Si dà vita, in questo modo, ad un processo positivo che può indurre i partiti più piccoli a ricondurre la loro funzione nell'ambito degli schieramenti più grandi, esprimendo e interpretando le nuove istanze popolari e quel dissenso che è vitale per la democrazia all'interno dei due schieramenti principali. Allora, anziché contestare l'accordo, si prenda l'occasione delle elezioni europee per dar vita ad una rinnovata espressione di partecipazione democratica. Vorrei ricordare un recentissimo sondaggio dell'IPSOS su questa materia e su questo disegno di legge: da esso emerge che il 70 per cento degli italiani è favorevole all'introduzione all'introduzione dello sbarramento del quattro per cento e che oltre il 40 per cento lo vorrebbe ancora più elevato. Ciò significa che i cittadini vogliono modernità, semplicità, ed assomigliare ogni giorno di più alle grandi democrazie europee alle quali oggi ci ispiriamo. Devo dire che per contrastare l'approvazione di questa legge elettorale si è fatto spesso ricorso ad argomenti discutibili e sproporzionati: si è tentato di demonizzare lo sbarramento del quattro per cento, cercando di stabilire confronti inaccettabili con la cosiddetta legge truffa di democristiana memoria, o addirittura con la legge Acerbo, che doveva servire a Mussolini per mettere fuori gioco il Parlamento italiano. Non si tiene conto che il ricorso allo sbarramento, con perfetto equilibrio delle forze politiche, in alternanza tra loro al governo del Paese, è funzionale alla creazione di un bipartitismo stabile e duraturo. Il ricorso a questa tecnica elettorale non avviene a discapito del nostro consolidamento democratico nel contesto europeo, ma, al contrario, serve al nostro Paese per recuperare quell'evoluzione democratica che i nostri partner europei e le più grandi Nazioni del mondo occidentale hanno avuto prima di noi. Se questo disegno di legge scaturisce da un'intesa politica tra l'attuale maggioranza e l'opposizione, ciò non può comportare l'implicito sospetto di un inconfessabile accordo sotterraneo. Al contrario, di fronte ad una politica come la nostra, l'intesa sulla nuova legge elettorale per le elezioni europee dovrebbe rappresentare una pietra miliare nella costruzione della democrazia italiana: sarà lo strumento tecnico e legislativo che potrà conferire nuova stabilità politica al nostro sistema. Il valore del bipartitismo oggi in Italia e in Europa è soprattutto quello di conferire stabilità politica alla moderna democrazia, di garantire l'espressione del consenso popolare, senza minimizzare il dissenso, che può oscillare, una volta a destra e una a sinistra, in occasione delle consultazioni elettorali. Con questa premessa, ci accingiamo ad affrontare le elezioni europee, consapevoli anche delle lacune istituzionali e dei ritardi dovuti ad una transizione interminabile, ma decisi ad imprimere una forte accelerazione al nostro sistema politico. Passando ora alla questione della rappresentanza femminile; con la senatrice Leddi abbiamo presentato un emendamento

una modifica predisposta al fine di dare copertura costituzionale a tutti quei provvedimenti legislativi ed amministrativi con i quali si volessero garantire forme di paritaria partecipazione tra donne e uomini, in particolare nella designazione di cariche elettive. Successivamente, nel 2004, con il ministro Prestigiacomo è stata introdotta nella legge elettorale per le elezioni europee una norma di garanzia del 30 per cento a favore del sesso meno rappresentato nelle liste elettorali, a pena di sanzione finanziaria per le formazioni politiche inadempienti. Nonostante ciò, attualmente l'Italia è al ventiduesimo posto in Europa per numero di donne elette al Parlamento europeo con una percentuale pari al 19,2 per cento. Dunque, esiste ben evidente una situazione di sottorappresentazione politica femminile. Se, infatti, l'attuale legge per le elezioni nazionali introducendo le liste bloccate ha di fatto permesso di aumentare decisamente la rappresentanza femminile all'interno del Parlamento italiano, ciò non è avvenuto con le elezioni europee. L'idea forte di un riequilibrio rappresenta quindi un elemento di qualità e di compiutezza del sistema democratico, ponendo termine ad un'anomalia della società italiana, dove le donne si affermano assumendo ruoli di responsabilità sempre maggiori ma continuano ad essere estranee alle assemblee elettive. Abbiamo migliorato, ma non dobbiamo abbassare la guardia su questo argomento e spetta, a mio giudizio, proprio a noi donne, e proprio in queste Aula, tenerlo alto. Dobbiamo farlo tutte insieme, perché è evidente che è un tema trasversale sul quale c'è un ampio consenso visto che quando si parla di pari opportunità si parla ormai di diritti civili e di libertà individuali.

e donne. Mi piace ricordare, in conclusione, un passo tratto dalla Repubblica di Platone, dove è scritto che non c'è un'occupazione che sia propria di una donna in quanto donna né di un uomo in quanto uomo, perché le attitudini naturali sono parimenti conferite ad entrambi e natura vuole

rispetto alla scorsa legislatura si sono ridotti da 14 a sei: a questo noi dobbiamo puntare anche nel nuovo Parlamento europeo.

per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, si individuarono alcuni problemi e alcune questioni da risolvere. Non si poterono risolvere in quella circostanza e si auspicò di ritornare sull'argomento negli anni seguenti, prima delle successive elezioni europee, che si svolgeranno tra pochi mesi. Le vicende politiche e parlamentari di quei cinque anni hanno

in questo breve periodo della legislatura in corso, è stato possibile solo questo intervento, un intervento importante sul quale si è concentrata l'attività

andranno riesaminati e io spero che nei prossimi anni vi sia davvero la possibilità di affrontare in modo efficace, ad esempio, il problema dello slittamento dei seggi dalle circoscrizioni più piccole

le liste bloccate sono quelle attraverso le quali quasi tutti gli altri Paesi europei eleggeranno i loro rappresentanti al Parlamento europeo. Noi li eleggeremo sulla base delle

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

della discussione generale, come Repubblicani europei abbiamo presentato degli emendamenti e siamo fermamente contrari a questa modifica del testo di legge che regola le elezioni dei deputati italiani al Parlamento europeo. Lo siamo con convinzione perché riteniamo che una riforma di questa legge elettorale avrebbe dovuto prevedere più incisivi accorgimenti democratici e, soprattutto, avrebbe avuto bisogno di un consenso popolare acquisito non *ex post*, ma *ex ante.* presupporre un dibattito che all'interno degli stessi Gruppi parlamentari doveva essere centrato sulla qualità delle riforme che si proponevano in funzione di un progetto di Europa, di quella Europa che vogliamo, di quella Europa politica che stenta a realizzarsi, che stenta ad alzare il alzare il capo a fronte di una politica globale dentro la quale conta poca o nulla, perché non compete come Continente, ma con le volontà di singoli Stati che, di volta in volta, si affacciano con prepotenza sulla scena politica mondiale dicendo la loro in maniera spesso scoordinata. È un dato di fatto che abbiamo sotto gli occhi tutti quanti ogni giorno e che avrebbe dovuto indurre ad un comportamento più serio da ambo le parti. sia stata una volontà di vertice da parte del centrodestra e del centrosinistra che ha portato, per altri fini e per altri obiettivi, ad una riforma che riguarda soltanto la soglia e che penalizza le le voci alternative, le voci originali che attraverso una cultura storica si sono sempre cimentate a livello democratico nel nostro Paese combattendo le più grandi battaglie per la democrazia

tanto nel centrodestra, quanto nel centrosinistra che la mia cultura laica e libertaria mi consente di rifiutare totalmente. Non è possibile accettare una volontà così marcatamente antidemocratica qual è quella che ha espresso questa riforma con l'introduzione di una soglia di sbarramento che

Stiamo discutendo della riforma di una legge elettorale; stiamo discutendo di regole e credo che quantomeno quando si parla di regole una maggiore attenzione dovrebbe essere meritata da parte di tutti noi. SBARBATI *(PD)*. La ringrazio per la sua fine cortesia, Presidente. Riprendendo il discorso poco fa interrotto, dicevo che non è possibile pensare che tutte le volte ci si scalda l'animo

le voci minoritarie, che spesso sono voci singolari anche con particolari caratteristiche dal punto di vista storico e culturale, siano il sale della democrazia, perché spesso portano avanti un pensiero divergente che non è un pensiero antagonista, ma è un pensiero su cui si può discutere democraticamente facendo un confronto culturalmente alto ed elevato per trovare le soluzioni migliori. Se ci impediamo questo tipo di confronto perché vogliamo comunque la *reductio ad unum*, sparizione dei piccoli partiti, quelli che qualcuno definisce con sprezzante ironia quelli dello 0,5 per cento. L'ho detto prima e lo ripeto, Presidente: sono contenta di essere uno 0,5 per cento, perché non ho mai venduto la mia storia, non ho mai venduto la mia cultura a nessuno. Ho fatto alleanze, ma sono rimasta quella che ero; sono repubblicana,

e solleticante - da un certo punto di vista - derisione, che in questo Parlamento si può avere di fronte alle mie parole. Le dico con fermezza, le dico con orgoglio, le dico anche con la coscienza che probabilmente non sortiranno alcun effetto, perché le decisioni sono state già prese;

le circoscrizioni elettorali del Lussemburgo sono ben diverse da quelle dell'Italia; 15 milioni di persone votano in una nostra circoscrizione e 40.000 persone votano in una circoscrizione lussemburghese. Quando si parla di Europa bisogna sapere cosa si dice; bisogna esserci stati e capire. Io sono stata nove anni nel Parlamento europeo e so di cosa parlo.

i partiti cosiddetti più grandi sono quelli che hanno il maggior numero di assenze rispetto a quelli che hanno magari un solo rappresentante o sono molto più piccoli. Questo a garanzia della rappresentatività degli interessi del nostro Paese e di un concetto di Europa all'interno di quel Parlamento che noi vogliamo o diciamo di voler difendere. Quindi, il mio voto è a favore degli emendamenti presentati e li sostengo assieme a chi la pensa come me. *(Congratulazioni)*.

La *ratio* di questo emendamento è piuttosto evidente, vale a dire la necessità, a causa dell'approssimarsi della scadenza elettorale, di ridurre il numero delle firme necessarie per poter presentare delle liste. È del tutto evidente che in un'altra contingenza, cioè qualche mese fa, questa stessa normativa avrebbe avuto una prosecuzione più ovvia poi nella pratica. A ridosso del voto, evidentemente, chi intende presentarsi, avendo come base di riferimento la precedente normativa, non ha più il tempo tecnico per potersi attrezzare e raccogliere le firme dovute.

ho contestato anch'io la lettura dell'articolo 97 per cui l'emendamento 1.101 è stato ritenuto improponibile, perché non ritengo che esso verta su La nostra discussione è sulla legge elettorale europea nel suo complesso e deriva da nove disegni di legge presentati alla Camera, ridotti certamente ad un intervento chirurgico dall'approvazione della Camera cioè la decisione in sequenza oggettiva a quanto stabilito dalla Camera dei deputati, se vogliamo lo introduciamo con norma costituzionale e non per prassi regolamentare con interpretazioni così restrittive come quella che abbiamo visto questa sera. L'emendamento riguarda la disarticolazione della circoscrizione isole per le elezioni europee. Mi rifaccio all'argomento della discussione generale: non è possibile sganciare completamente da un rapporto reale tra un territorio realmente isolato, realmente diverso da quello al quale è artificialmente collegato, il tema della rappresentanza politica nel Parlamento europeo. La devitalizzazione di questa rappresentanza ha comportato per la Sardegna 15 anni di difficoltà e di negazione di rappresentanza nel Parlamento europeo. Io ne prevedo altri cinque, per arrivare complessivamente a venti. Non basta dire che siamo pronti a discutere di questo tema dopo le elezioni europee. Bisognava farlo adesso. Registro, e voglio dire a questa Camera, che tra gli impegni presi

collega Germontani e che credo sarà sottolineato da altri interventi che seguiranno, cioè quello della rappresentanza femminile. Sembra che in questo Paese si sia dimenticato che l'articolo 51 della Costituzione ha cambiato anche i parametri cui dovrebbero attenersi le leggi elettorali. Anzi, sembra che questo sia quasi un elemento da derubricare dagli accordi politici e dalle Aule parlamentari. Credo che sia stato davvero un grave errore non aver pensato che in questa occasione si potesse dare un segnale, come Paese - ripeto come Paese non come schieramento politico o come Governo di essere almeno verosimilmente un po' più vicini agli altri Paesi europei, ai nostri partner europei. Noi non solo siamo indietro rispetto all'Europa. Siamo indietro rispetto a moltissimi Paesi in via di sviluppo e a moltissimi paesi che hanno raggiunto molto più tardi noi le soglie della democrazia parlamentare. I dati della rappresentanza italiana per quanto riguarda le donne nelle Assemblee elettive sono davvero molto bassi;

abbiamo visto che quando le donne sono impegnate, soprattutto nelle amministrazioni locali, esse sanno farsi interpreti di una politica più vicina alle persone e più aderente alle persone e più aderente alla realtà. Credo che anche questo sia un contributo di innovazione e qualità alla politica stessa. C'è poi una questione profondamente democratica,

con gli emendamenti sull'ammissibilità delle liste, sia su quelli della preferenza di genere, fare un passo avanti in questa direzione: è stata un'occasione mancata, ed è stata un'occasione mancata anche non poterne discutere in quest'Aula e verificare la convergenza, che credo ci sarebbe stata, di altre parlamentari e parlamentari sulla questione.

che non ha funzionato quello che è stato fatto finora: la delegazione italiana al Parlamento europeo è composta da 78 parlamentari; le donne sono soltanto 16, cioè il 12 per cento, e voglio aggiungere che molte di queste donne sono entrate grazie al fatto che alcuni uomini si sono dimessi, quindi in prima elezione erano state escluse. Dunque portiamo la maglia nera Abbiamo cambiato la Costituzione aggiungendo un comma all'articolo 51, proprio per dare copertura costituzionale a leggi che prevedessero misure a sostegno delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle istituzioni: poco e niente è successo. Sono difficili i cambiamenti in questo settore e lo sappiamo tutti. La cittadella della politica è difficilmente espugnabile da parte delle donne: voglio usare questa immagine militare che non mi si addice, ma che corrisponde alla realtà. Ma perché questo? Lo voglio chiedere e ne voglio discutere interloquendo anche con i colleghi rappresentanti del genere maschile: perché tanta resistenza ad adottare misure che introducano reali pari opportunità tra uomini e donne nella rappresentanza istituzionale? La risposta non è difficile; qui c'è un conflitto oggettivo: conflitto oggettivo: se una donna viene eletta, un uomo deve andare a casa. Ma è anche perché la politica rappresenta ancora il luogo del potere per eccellenza, il luogo in cui si stabiliscono le regole e si può stabilire anche la regola di escludere, come quella che abbiamo discusso in occasione della legge sulle quote, quando il centrodestra ha cambiato la legge per il Parlamento nazionale.

la democrazia paritaria esige, richiede, la partecipazione di donne e uomini alla costruzione delle sue istituzioni; richiede una condivisione dello spazio pubblico e una eguale responsabilità degli uomini e delle donne. Siamo convinti e convinte che una democrazia paritaria sia più ricca, più piena e più coesa.

dell'emendamento 1.104 consiste nel volere dare uno strumento in più per fare un passo avanti verso questa democrazia paritaria.

come potrebbe essere, ad esempio, l'inammissibilità della lista che non rispetta le leggi - ha portato a 16 parlamentari elette su 78. Diciamo, allora, che non ha funzionato e che se vogliamo davvero risolvere questo problema e lo abbiamo a cuore dobbiamo introdurre norme diverse. La norma che noi proponiamo ‑ e concludo ‑ è prevedere che sia obbligatorio

esclusa. Non è un rivendicazionismo corporativo perché noi mettiamo al centro la qualità della nostra democrazia e della sua capacità di rappresentanza. Noi vogliamo costruire una democrazia più moderna, capace di tener conto anche dei desideri di rappresentanza e di protagonismo delle donne. Mi dispiace che questo dichiarato improponibile. Mi auguro che questa Aula, per iniziativa delle parlamentari e dei parlamentari, possa in un altro momento discutere e prendere in considerazione una proposta di legge che preveda questo. *(Applausi

sulla decisione di considerare improponibile l'emendamento 1.106. Presidente, comprendo che questo è un provvedimento blindato, ma se non in questa sede in quale sede si pone rimedio a

inadeguata perché risolve un problema. Il tema delle circoscrizioni per le elezioni europee, nella loro ingestibilità politica sul piano del rapporto eletto/elettore, è sotto gli occhi di tutti. Il tema delle preferenze, che a noi è tanto caro, insieme a quello delle spese relative alla campagna elettorale diventano dei problemi politici seri con circoscrizioni così ampie. Non è assicurato alcun collegamento tra eletto ed elettore e si impongono spese elettorali eccessive che o

democrazia chiarissimo: dobbiamo costruire soluzioni che siano razionali e garantiscano la rappresentanza. Signor Presidente, credo che consentire il voto di questo emendamento sarebbe stato un atto chiaro di assunzione di responsabilità con cui i miei colleghi parlamentari, per quanto vincolati alle regole di partito, potevano esprimere un'opinione che poteva essere importante simbolicamente. Anche se non avesse raggiunto la maggioranza dei consensi di questa Aula, era un'occasione per porre questo tema al centro del dibattito politico.

la Presidenza è stata estremamente rigorosa, anche per una motivazione che probabilmente molti non conoscono. deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato di porre all'ordine del giorno, sostanzialmente operando uno stralcio, il semplice articolo che riguardava la soglia di sbarramento del sistema elettorale europeo.

che la Camera possa espungerle nuovamente in quanto fuori dal deliberato di quella Conferenza dei Capigruppo. Nella logica e nella sinergia di un leale rapporto di collaborazione tra Camera e Senato e nella logica della buona legiferazione e della gestione del processo legislativo, questa Presidenza non poteva ignorare quel deliberato, che - ripeto e concludo - concentrava la propria attenzione sull'esigenza e sull'inderogabilità di dare attenzione e priorità soltanto al tema della soglia.

Mi sembrava doveroso dare questa spiegazione ai colleghi perché avevano il diritto ad una motivazione aggiuntiva rispetto alla semplice dichiarazione di estraneità di materia. Ciò detto,

intervengo molto brevemente comprendendo perfettamente lo spirito della decisione della Presidenza del Senato. Con l'emendamento 1.0.100 abbiamo voluto segnalare ai colleghi l'opportunità di rivedere il divieto del terzo mandato consecutivo dei sindaci limitatamente ai piccoli Comuni. Naturalmente per i Comuni di maggiori dimensioni il problema assume delle valenze delle valenze e dei significati particolari e su questo vi sono opinioni molto diverse. Per quanto riguarda i Comuni sotto i 5.000 abitanti, il problema si pone invece con una peculiarità che va considerata.

le piccole comunità insistono perché un buon sindaco possa restare ad espletare quel ruolo anche oltre il secondo mandato. L'esigenza è ampiamente condivisa e il ministro Maroni, nel corso di un'audizione in Commissione affari costituzionali,

BONINO *(PD).* Signor Presidente, colleghi, interverrò sull'insieme degli emendamenti, annunciando che la delegazione radicale li sosterrà quasi tutti. sia consentito di motivare brevemente la ragione. Onorevoli colleghi, voi potete ammantare questa legge di grandi e nobili motivazioni, ma ciò che è indubbio è che essa risponde a convenienze italiane, di tutti i partiti politici qui rappresentati, dei maggiori, dei due più grandi, dell'Italia dei Valori e dell'UDC,

Dico questo perché non mi iscrivo tra coloro che pensano che mettere uno sbarramento del 4 per cento sia un attentato alla democrazia; né penso e pensiamo noi radicali che la reintroduzione delle preferenze sia di per sé un dato di democrazia. Sono parlamentare di lungo corso e so come funzionano e come funzionavano le preferenze. So perfettamente che non è così. Le preferenze funzionano o per censo o per cordata o anche per voto di scambio, quindi non mi inserisco in questo dibattito. Mi inserisco invece su una questione ben più grave. più grave. Non è che questa legge ammazzi la democrazia: noi riteniamo che lo Stato di diritto nel nostro Paese sia da lungo tempo moribondo, se per Stato di diritto si intende quel sistema che ha la certezza delle regole, i paletti, i limiti e tutti gli istituti di controllo funzionanti. Questo nel nostro Paese non c'è più da tanto tempo e penso quindi che si fanno prevalere convenienze ed espedienti di brevissimo respiro, francamente. La debolezza italiana nelle istituzioni europee - fatevelo dire da chi le ha frequentate da tanto tempo - non è dovuta alla frammentazione, si fa per dire, della delegazione italiana al Parlamento europeo, bensì ad altre e più profonde ragioni, ivi compreso il fatto che poco ci vanno i nostri parlamentari, poco ci sono e poco si fanno sentire. Nella nostra e vostra

la situazione e lo stato dell'arte dell'Europa in generale non è brillante, e quanto ne avremmo bisogno in questo momento di crisi economica! di questa legge, che è solo un ulteriore colpo rispetto a una situazione in cui la certezza delle regole non c'è nel nostro Paese, a partire dalla certezza della pena. Continuiamo e continuate a funzionare per leggi e leggine di emergenza. Soprattutto, voglio ricordare che c'è una regola base della democrazia, di stampo degasperiano e quindi certamente non estremista, che è il conoscere per deliberare. In questo Paese l'utilizzo spesso consociativo degli strumenti di informazione, pubblici e privati, fa sì che l'espulsione di forze politiche e di temi dall'agenda dei *media* italiani ha raggiunto livelli che dovrebbero preoccupare non solo noi, ma penso tutti e anche tutti voi. Conoscere per deliberare non è dato e dispiace che forze politiche, che oggi urlano al golpe per l'introduzione dello sbarramento del 4 per cento, di tutti questi processi non si siano mai occupati. Spiace altresì che non ci siano i paletti che fanno sì, come in altri Paesi, che il potere non sia senza freni e senza inibizioni, e che la maggioranza sia forte non solo dei numeri, ma quando rispetta le regole che si è data. Questo non avviene più e, badate, credo che gli esempi di questi ultimi giorni, in tema elettorale e non solo, dovrebbero preoccupare molti, perché la politica è quella cosa fragile in cui la ruota gira. gira. Ciò che ci dovrebbe accomunare è esattamente il rispetto verso l'opinione pubblica, che deve essere messa in condizione di scegliere e non di essere scelta, perché essa perché essa si forma sul contraddittorio, non sul lavaggio del cervello. Questo può funzionare e funziona ovviamente, ma ha il respiro molto corto.

di uno slabbramento delle regole democratiche del nostro Paese, che non nasce oggi ma viene da molto più lontano. Avete bloccato per mesi, insieme, la Commissione di vigilanza

non avranno effetto su una RAI lottizzata e che vi apprestate a rilottizzare tranquillamente mercoledì sera. Tutto questo ci pone ad essere francamente alternativi a questo modo di procedere ed al modo di considerare le leggi elettorali ed i cambiamenti delle stesse come espedienti di convenienza immediata, che poco hanno a che vedere rispetto a quella che dovrebbe essere essere l'unica riforma seria che dovremmo fare: il sistema uninominale a collegi piccoli, in cui i candidati sono conosciuti da tutti e

quando non rivoltante, di accordi più o meno inaccettabili. Per questi motivi sosterremo quasi tutti gli emendamenti, ma vi diciamo anche che non è la vittoria di un giorno, di un momento, di uno spezzone di legge che può rendere più forti le istituzioni del nostro Paese. Al contrario!

Mi permetto, tuttavia, di osservare che la sacrosanta esigenza di armonizzare i lavori tra le due Camere non si può spingere fino al punto di soffocare l'essenza stessa del bicameralismo ammutolendo di fatto uno dei due rami del Parlamento. dei senatori Sanna, Passoni ed altri fosse stato, come mi auguravo, ammesso, ne avrei chiesto la votazione per parti separate, con particolare riferimento alla lettera *a),* che prevede la suddivisione della circoscrizione insulare nelle due parti principali dell'isola di Sardegna e dell'isola di Sicilia. Ciò a motivo del fatto che, come è noto, a causa della sproporzione di popolazione esistente tra le due isole, da 15 anni alla Sardegna non è consentito di esprimere un rappresentante nel Parlamento europeo. Mi permetto di ricordare che da almeno tre secoli, tutte le leggi elettorali hanno fatto valere quello che nella tradizione anglosassone si chiama il naturale interesse del candidato a rappresentare il proprio territorio. Questo naturale interesse è tanto più accentuato quando si tratti di un territorio così nettamente definito come quello di un'isola. Nei fatti, la norma elettorale ora in vigore nega ai sardi non teoricamente, ma di fatto la possibilità di rappresentare la Sardegna nel Parlamento europeo.